Presidente, desideravo complimentarmi con il senatore segretario Eufemi per come ha letto il verbale. Sono riuscito a capire tutto quello che ha detto. Non così è successo altre volte e credo che sia una mancanza intollerabile perché questo è l'unico momento in cui possiamo

che mi pare stia emergendo nel rapporto tra i lavori del Senato e quelli della Camera a proposito del Documento di programmazione economico-finanziaria. Naturalmente non sta a me deliberare, non sta a me deliberare, ma credo sia mio dovere segnalare, sia a nome della maggioranza della Commissione bilancio sia - credo - a nome dell'opposizione, che si sta determinando sui lavori relativi al Documento di programmazione economico-finanziaria un problema

presentano risoluzioni; queste sono di particolare rilievo perché in rapporto alle scelte compiute dal Governo con il DPEF definiscono definiscono le proposte di politica economica e sociale che la maggioranza e l'opposizione intendono perseguire negli anni successivi. I colleghi sanno che proprio per questo è assolutamente ragionevole - infatti è sempre accaduto - che le risoluzioni presentate rispettivamente dalla maggioranza e dall'opposizione fossero tra

Si sta, invece, delineando, in base al calendario dei nostri lavori e dei lavori della Camera, una situazione nella quale la Camera voterebbe le risoluzioni sul DPEF - non mi riferisco alla discussione, ma al voto sulle risoluzioni - addirittura con sette o di differenza. Risultando chiaro che le risoluzioni devono essere se non identiche certamente sovrapponibili, si sta determinando una situazione nella quale i colleghi della Camera potrebbero ritenere in buona sostanza di non avere effettivamente avuto e di non avere, almeno formalmente, spazio adeguato per influire sulla determinazione dei contenuti delle risoluzioni approvative del DPEF o, nel caso nel caso dell'opposizione, di contrapposizione alle scelte del DPEF, determinando una situazione che sia per la maggioranza che per l'opposizione come minimo potrebbe essere definita antipatica sul piano istituzionale. È per questa ragione che volevo evidenziare - so che è del tutto inappropriato in rapporto alle prerogative della Conferenza dei Capigruppo, che ha stabilito l'ordine delle votazioni, il nostro ordine del giorno, il calendario e così via e così via - come, secondo me, si sta determinando una situazione nella quale nel rapporto tra Camera e Senato potrebbe insorgere un vero problema istituzionale; non dico un conflitto ma qualcosa di molto simile. allora rivolgere a lei e, tramite lei, al Presidente del Senato, per valutare se non sia preferibile una piccolissima variazione del calendario, al fine di consentire che la votazione delle risoluzioni sul quella - avvenga, per esempio, martedì mattina prossimo e non nella giornata di domani. Se avverrà infatti nella giornata di domani ciò significa che i colleghi della Camera dovranno votare quelle stesse risoluzioni, o risoluzioni sostanzialmente analoghe,

Credo che la Camera voterà nella giornata di lunedì il DPEF, quindi lo spazio intercorso sarà di tre giorni. La situazione che si è verificata non dipende da un mancato accordo Camera-Senato, ma dal fatto che questa settimana la Camera approverà il decreto-legge sul cosiddetto "tesorotto" - per dirla come il

È sempre successo nel passato che un ramo del Parlamento approvasse delle risoluzioni anche a una settimana di distanza, quindi non c'è niente di nuovo. In realtà, credo che tutto il problema sia dovuto al fato che la maggioranza non sa cosa vuole scrivere nella sua risoluzione; ma allora il Senato non deve fare da levatrice all'incapacità della maggioranza di coordinare se

Nella Conferenza dei Capigruppo di ieri, lo dico per i colleghi che possono non saperlo, si è lungamente discusso, come credo il presidente Calderoli sa, proprio dei lavori parlamentari del Senato di questa settimana e della settimana prossima e si è valutata la possibilità in cui il DPEF venisse votato dalle due Camere a tre giorni di distanza l'una dall'altra. Si è però considerato che era l'unico modo per consentire al Senato di approvare il cosiddetto decreto‑legge sul tesoretto la settimana prossima. È ovvio che se la maggioranza tutta dovesse dire che il decreto-legge sul tesoretto viene abbandonato, la settimana prossima potremmo votare il DPEF. Scelga la maggioranza. Ieri la maggioranza ha scelto di votare il DPEF questa settimana e il decreto‑legge sul

che abbiamo appreso dai giornali di oggi che ieri il Presidente del Consiglio avrebbe in qualche modo trovato il modo di far stanziare 1,5 miliardi di euro per opere pubbliche in Sicilia e casualmente è mancato il senatore del Movimento popolare per le Autonomie. Non avanzo sospetti, mi limito a constatare che c'è stata una sorta di dare-avere. La battaglia per la Sicilia e per il Mezzogiorno noi non l'abbiamo mai ridotta a mercanteggiamenti: voti in Senato di questo o quel senatore. Sono battaglie politiche e strategiche come quelle che la Lega fa per le Regioni del Nord; noi intendiamo che queste due battaglie siano coordinate per un'unità nazionale diversa. Mi limito a rilevare che il Presidente del Consiglio ha ritenuto di dare 1 miliardo e mezzo di euro per le opere pubbliche in Sicilia casualmente il giorno in cui il senatore del Movimento popolare per le Autonomie era assente. È una cosa strana, mi limito a rilevare questa stranezza, Presidente.

Signor Presidente, questo disegno di legge rappresenta sicuramente un fatto positivo per l'organizzazione dei Servizi di sicurezza e soprattutto, ciò che più conta, per la sicurezza dello Stato. Ci sono diversi elementi che innovano la realtà dei Servizi di sicurezza e la adeguano alla situazione che indubbiamente è molto mutata da quando nel 1981 fu votata la legge fino ad oggi in vigore. In particolare possiamo citare tra i fatti positivi una divisione chiara e razionale tra le competenze dei due Servizi. Oggi le competenze sono difficili da individuare e dunque anche le responsabilità. La divisione tra sicurezza esterna e sicurezza interna risponde alle esigenze dei nostri giorni, dei nostri anni, e consente una più facile individuazione delle rispettive competenze e dunque delle rispettive responsabilità. Positiva anche la riconduzione al Presidente del Consiglio della responsabilità dei Servizi nel loro insieme.

perché non appare, quantomeno al momento, così chiara la divisione di compiti tra di essi. Io conto che nel prosieguo del dibattito questo emerga ed eventualmente possano essere individuate misure per chiarificare anche nel testo queste eventuali incertezze. È anche estremamente importante che si siano definite in modo chiaro, anche con l'introduzione di alcuni nuovi articoli nel codice

abbiano la possibilità di svolgere il loro difficile lavoro nel modo migliore, coperti da garanzie che devono, giustamente, avere limiti rigorosi - e limiti rigorosi ci sono in modo che oltre ai rischi di carattere fisico che affrontano spesso, agendo in zone o in ambienti estremamente difficili ed estremamente pericolosi, abbiano anche un'adeguata tutela dal punto di vista legale. di elementi molto importanti, che però devono necessariamente essere accompagnati da una reale attuazione di ciò che anche in questo disegno di legge viene espresso esplicitamente ma che non deve passare in secondo piano per il solo fatto che è, di solito, contenuto nell'introduzione dei commi uno dei diversi articoli, e cioè il principio di leale e fattiva collaborazione tra i vari organi dello Stato, tra il Governo e i Servizi, naturalmente (poiché i Servizi dipendono dal Governo), l'attività svolta per la sicurezza dello Stato, la magistratura e, ovviamente, le forze dell'ordine. Questo il disegno di legge lo specifica e lo richiede; naturalmente poi però le le leggi e le procedure vengono applicate da uomini e da donne e a loro dovrà essere richiesta una particolare attenzione, una particolare lealtà e spirito di collaborazione che non deve cedere a esigenze di altro tipo, a esigenze di carattere politico o, peggio ancora, di carattere mediatico.

dei Servizi segreti che hanno prestato e prestano la loro opera al servizio dello Stato vengono dati in pasto ai *media* attraverso operazioni giudiziarie quantomeno spericolate.

altresì, che la legge oggi in vigore fu un passo avanti all'epoca perché delineò le procedure precise che dovevano essere seguite quando ai Servizi segreti giungevano informazioni

si è ritenuto, dal momento che la questione è stata fatta emergere da una Commissione non gradita all'attuale maggioranza di Governo, di trascurare, di trascurare, ignorare o addirittura negare quanto è emerso in modo molto chiaro ed è stato peraltro riportato alla magistratura.

agiscono sotto i riflettori televisivi, anzi i loro successi maggiori sono quelli che non vengono neppure conosciuti dall'opinione pubblica. Quando negli scorsi anni anni sono stati arrestati gruppi e persone che avevano l'intenzione di compiere attentati terroristici nel nostro Paese - come ne sono stati compiuti in altri Paesi in questi anni -, ebbene, queste notizie logicamente notizie logicamente non hanno avuto grande rilievo sui *media*, ma si sono rivelate importantissime: se non fossero avvenuti quegli arresti, avremmo avuto notizie di molto di molto maggior rilievo e, soprattutto, molto più tragiche. Avremmo avuto notizia di attentati, di decine o centinaia di morti, com'è avvenuto in altri Paesi.

Sappiamo anche che l'uomo che morì nel portare a compimento la liberazione di uno di questi ostaggi apparteneva a questi Servizi. Dobbiamo per gratitudine a lui e ai tanti uomini e donne che lavorano in questi settori essere essere spinti a un senso di responsabilità nell'applicare le leggi. In questi giorni, in questa mattinata, il senso di responsabilità si applica nell'approvare una legge certamente migliorativa, che consentirà a chi lavora per la sicurezza dello Stato (cioè dei cittadini) di operare con più serenità, pur svolgendo un compito estremamente difficile, spesso disconosciuto, e a volte addirittura perseguito per via giudiziaria.

e all'acquisizione di notizie in qualsiasi modo rilevanti per la difesa della propria integrità e della sicurezza pubblica. La cultura giuridica italiana ha affrontato più volte il problema della definizione di questo diritto ed ha analizzato le norme e le strutture istituzionali che ad esso fanno capo, anche in tempi nei quali la materia dell'*intelligence* non aveva una regolamentazione legislativa certa e compiuta. Un lucido inquadramento teorico di questo diritto all'informazione dello Stato democratico si trova già in un saggio di Arturo Carlo Jemolo, pubblicato nel 1967, volto a richiamare l'attenzione dei costituzionalisti su un aspetto trascurato della struttura statale, ma presente ed attivo. Numerosi spunti offerti dal saggio sono stati poi ripresi dalla letteratura giuridica, in specie quegli aspetti nei quali si prospetta la necessità di nuove garanzie. Già nello scritto di Jemolo e poi nella dottrina successiva venivano fissati, nel definire il diritto di informazione e di prevenzione dello Stato, tre limiti necessari. Il primo,

da potenziali minacce all'integrità dello Stato: nemici esterni o nemici che, all'interno dei confini nazionali, rappresentano un pericolo concreto per la vita democratica del Paese e per la sicurezza dei cittadini. Il secondo limite è che la raccolta di informazioni sulle idee politiche dei cittadini è illegittima e tutto ciò che ha a che fare con la libera manifestazione del pensiero, con la libertà di movimento, con l'esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti non può essere in alcun modo oggetto di una raccolta di informazioni riservate.

nell'attività dei Servizi di informazione e sicurezza. Per deviazioni intendo tutti i comportamenti in contrasto con i princìpi della Costituzione e con il dovere di legittimità, cioè di rispetto delle regole finalizzate all'esercizio dell'attività di prevenzione e raccolta di informazioni riservate per la tutela dell'integrità dello Stato e non di interessi particolari. Cari colleghi, da questi princìpi ancora oggi validi discende, a mio giudizio, un dovere specifico, che è proprio dei Servizi di informazione e sicurezza: vi sono informazioni, vi sono *dossier* che riguardano l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, che riguardano l'esercizio della libertà delle persone e dei cittadini, che non possono formare oggetto dell'attività di *intelligence,* se esistono documenti che contengono informazioni di tal genere, questi documenti non possono essere conservati negli uffici pubblici dei Servizi di informazione e sicurezza, né possono far parte degli archivi delle strutture di *intelligence*. Bisogna intendersi su questo punto, perché questa è una discriminante che deve valere per tutte le attività dell'*intelligence*. cogente ed effettivo questo principio è necessaria una organizzazione certa e controllata degli uffici dei Servizi di informazione e sicurezza, dei loro archivi, della formazione e della conservazione dei documenti, e del controllo sul loro contenuto. Il disegno di legge che noi stiamo discutendo introduce novità rilevanti e significative: è, per la prima volta, una vera riforma. Noi abbiamo oggi una regolamentazione di questa materia che è fissata dalla legge n. 801 del 1977: quella legge appartiene ancora alla stagione della Guerra fredda. Tuttavia è stato il risultato di un impegno comune e di una collaborazione leale tra le forze politiche e parlamentari che la approvarono. Oggi è una legge datata, inadeguata e la sua inadeguatezza già si manifestò pochi anni dopo l'entrata in vigore, se è vero che proprio tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta noi abbiamo avuto alcune delle deviazioni più gravi tra quelle che si sono verificate nella storia dell'*intelligence* italiana. Si può dire che in quegli anni (che sono gli anni terribili della difficile lotta contro il terrorismo e sono tra l'altro gli anni dell'attacco al cuore della democrazia italiana, del sequestro e dell'assassinio di Aldo Moro) i Servizi di informazione e sicurezza nel loro insieme erano nelle mani della loggia massonica P2: il vero capo dei Servizi di informazione e sicurezza, tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, era Licio Gelli. Dunque quella legge, con il suo sistema di controlli, si è manifestata immediatamente, negli anni successivi alla sua approvazione, del tutto inadeguata. Come non ricordare, dopo la fine della guerra fredda, la spartizione illecita dei fondi riservati del SISDE? Anche là i controlli non funzionarono. Non credo di violare alcun segreto, poiché già questo questo dato è stato richiamato in una relazione del Comitato parlamentare dei Servizi: vi è un verbale del Comitato parlamentare che risale, se non ricordo male, alla fine degli anni Ottanta, nel quale, durante l'audizione del ministro dell'interno Antonio Gava, il presidente di quel Comitato (e va a suo onore ricordarlo), che era Mario Segni, comunicò sulla base di informazioni che a lui erano pervenute, che esisteva un problema serio nell'ambito del SISDE e che quel problema riguardava attività illecite, disinvolta utilizzazione dei fondi. Il presidente del Comitato parlamentare dei Servizi, segnalò allora quelle anomalie al Ministro dell'interno, ma la sua segnalazione non ebbe alcun seguito, non ebbe alcun seguito, anche per l'estrema limitatezza dei poteri del Comitato parlamentare di controllo. Questa limitatezza noi l'abbiamo vista anche in anni recenti, anche di fronte a vicende drammatiche, come quella del sequestro di un cittadino straniero, che era tra l'altro sottoposto ad indagini penali in Italia: un sequestro avvenuto clandestinamente e sul quale il Comitato parlamentare di controllo, negli anni passati, ha ricevuto informazioni lacunose e non rispondenti al vero dai responsabili dell'*intelligence* e dai responsabili della guida politica dei servizi. Il Comitato parlamentare troppo spesso non riesce ad accertare i fatti: non esercita e non può esercitare un potere penetrante di controllo, di acquisizione di documenti, e si riduce quindi a svolgere un'attività marginale di assunzione delle informazioni che graziosamente le strutture di *intelligence* vogliono concedergli. Questa legge deve introdurre un elemento di novità e di discontinuità rispetto alla prassi insoddisfacente che abbiamo vissuto negli anni passati. Il Comitato parlamentare di controllo in questi anni ha svolto una funzione vera, ha accertato fatti, ha individuato responsabilità, soltanto nella misura in cui è riuscito a costruire un circuito di controlli raccordandosi all'autorità giudiziaria che indagava sugli illeciti commessi nell'ambito della attività di *intelligence*; ma ciò non può bastare, deve esserci una fisiologica capacità, un potere ordinario di controllo del Comitato parlamentare sull'attività dei Servizi, con tutte le garanzie

per la riservatezza che circonda i suoi lavori e che va rispettata, deve poter intervenire, deve poter conoscere, deve poter esercitare un controllo almeno pari a quello che esercitano gli organi parlamentari nei principali ordinamenti democratici, dagli Stati Uniti al Sudafrica, allo Stato di Israele, ove esistono organi parlamentari di controllo che sono degni di questo nome. C'è nella legge in discussione una disciplina nuova e particolarmente rilevante di aspetti che sono essenziali, quali la distinzione delle funzioni tra le diverse branche dell'*intelligence*. C'è un mutamento grande, una svolta, perché il controspionaggio, che per la verità negli anni passati non ha dato buona prova e che era nell'ambito del SISMI, viene spostato al Servizio di informazione e sicurezza le cui competenze riguardano la minaccia interna, e ciò corrisponde ad una scelta logicamente accettabile e fondata. Altre norme di grande rilievo intervengono nella materia del segreto di Stato. Per la prima volta nell'ordinamento italiano, che era tra i pochi ordinamenti democratici - non so se l'unico - ad avere un segreto permanente ed eterno, si introduce la temporaneità del segreto, che è un criterio innovativo di grande portata e permette un controllo *ex post*, un controllo successivo, sui documenti, sull'operato dei Servizi. Naturalmente questo controllo successivo ha un senso se è garantita la conversazione dei documenti, se è garantita una disciplina certa e sicura degli archivi, della loro composizione, della loro conservazione, del controllo su di essi. Le innovazioni più rilevanti riguardano la materia del segreto sotto il profilo della tutela amministrativa del segreto. Esiste nell'ordinamento italiano l'Ufficio centrale per la sicurezza, che fa capo all'Autorità Nazionale per la Sicurezza, che è fuori da qualsiasi regolamentazione legislativa. Per la prima volta, in questa legge si dà una regolamentazione legislativa all'Ufficio Centrale per la Sicurezza, alla materia dei Nulla Osta di Segretezza, che sono abilitazioni concesse a quei dipendenti pubblici che debbano trattare, per l'esercizio delle loro funzioni, documenti classificati, oppure abilitazioni concesse alle imprese che hanno lavori in appalto per i quali si pongono particolari problemi di sicurezza. Da anni ho sostenuto la necessità di procedimentalizzare la concessione del NOS e di introdurre una norma molto semplice: c'è un ufficiale, c'è un dipendente pubblico che ha bisogno del NOS per un avanzamento di carriera, gli si comunica che su di lui verranno svolti accertamenti al fine di stabilire se vi sia una sua vulnerabilità, una sua inadeguatezza al conseguimento al conseguimento del livello di funzioni che lo abilita a trattare documenti o materie coperte da un vincolo di segretezza. Egli può rifiutarsi di andare

Questa è una norma garantista. Per anni la proposta di una norma di questo genere si è scontrata con un muro di indifferenza. Oggi, per la prima volta, questa procedimentalizzazione viene stabilita con legge, questa garanzia viene introdotta da una norma

Infine, è importante che in questo disegno di legge si rafforzino i poteri di controllo del Comitato parlamentare anche rispetto ad un'altra novità rilevante, che è quella delle cosiddette garanzie funzionali. Si stabilisce un procedimento per cui in relazione a determinate condotte che comportano una violazione della legge di non grave portata, che non colpisce beni primari, interviene

degli appartenenti ai Servizi di informazione e sicurezza, il vertice dell'*intelligence*, e per esso poi il Presidente del Consiglio, si avvale dello strumento del segreto di Stato; strumento improprio, che alla fine copre tutto e che non offre le garanzie determinate invece

in base alla quale il Presidente del Consiglio, trenta giorni dopo la conclusione dell'operazione nell'ambito della quale sono state poste in essere condotte per le quali egli ha stabilito una causa di giustificazione, e ha dato la sua autorizzazione,

il cui svelamento potrebbe nuocere alla sicurezza dello Stato. Si tratta, colleghi, di norme di grande rilievo, conferiscono certezza all'organizzazione dell'*intelligence*, rendendo più autorevole il nostro sistema di *intelligence* anche nei rapporti con i Paesi amici, con quelli con i quali l'*intelligen**ce* italiana ha rapporti di collaborazione pressoché quotidiani. In passato l'organizzazione dei Servizi, e in particolare l'organizzazione addetta al segreto, erano disciplinate da norme regolamentari riservate. Esse facevano riferimento in modo diretto ad accordi tra le *intelligence* di Paesi alleati e segnatamente ad accordi - come il *Minimum standards of security* dell'inizio degli anni cinquanta - con l'*intelligence* statunitense. Oggi, per la prima volta a tanti anni di distanza dalla fine della guerra fredda, interviene una legge certa, conoscibile, compiuta, che regola l'intera materia e che quindi dà più forza, più autonomia più autorevolezza ad un'istituzione così importante come l'*intelligence* italiana nei rapporti con i Paesi amici e con le *intelligence* di quei Paesi. Dunque, la mia è una valutazione positiva su queste norme.

Un'*intelligence* che sia sottoposta ad un controllo certo e penetrante per ciò stesso viene legittimata e diventa più credibile agli occhi dei cittadini e sulla scena internazionale.

chiaramente anche all'organizzazione che si è dato di recente un Paese importante come gli Stati Uniti d'America, che ha voluto al vertice dell'organizzazione amministrativa un responsabile politico di quel Paese.

Per tale motivo abbiamo svolto un lavoro emendativo molto selettivo e delimitato e abbiamo deciso di non prendere in esame proposte che riguardassero sistemi del tutto differenti da quelli licenziati dalla Camera Pertanto, signor Presidente, colleghi senatori, abbiamo ritenuto che le proposte formulate dal senatore Ramponi non potessero essere accolte. Ciò, però, non significa che non abbiamo apprezzato quelle proposte, che sono tutte di grandissimo valore ed assolutamente interessanti.

ma anche perché avrei potuto e voluto apprezzare il lavoro emendativo da lui svolto, ma le condizioni politiche nelle quali si sono determinate quelle considerazioni non ce lo hanno consentito e penso di poter parlare anche a nome del correlatore, collega Pastore. Signor Presidente,

la parola "già". Il testo del dispositivo reciterebbe quindi: «impegna il Governo a garantire adeguate risorse per il funzionamento dei Servizi di informazione e di sicurezza già nel Documento di programmazione economico-finanziaria, in vista della predisposizione della legge finanziaria per il 2008».

per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo. Esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 21.17, 21.12, 1.200, 1.201, 6.200 e 7.200. Esprime parere di semplice contrarietà

che il sistema di sicurezza è costituito dal Presidente del Consiglio, dal Sottosegretario nominato e dal Dipartimento, che comprende anche le due Agenzie, a differenza di quanto dica la legge, non vi è assolutamente nessuna differenza. Pazienza: io ho condotto la mia battaglia, ho insistito all'infinito, ma non posso continuare. D'altra parte, il nostro è un rapporto fra gentiluomini che intendo mantenere.

comunque un'Autorità politica al vertice delle responsabilità dei Servizi, considerando che il Presidente del Consiglio non può dedicarsi continuamente a questo compito. D'altra parte, aspetto che il sottosegretario Micheli concluda la sua telefonata

«il Presidente del Consiglio nominerà un Sottosegretario addetto ai servizi» sia concetto improponibile,

nulla del sistema che voi avete concepito e che io accetto, perché, come ho già detto ieri, riprende moltissima parte del contenuto del disegno di legge iniziale.

la responsabilità della guida, del controllo? Anche i capi delle due agenzie si sentiranno molto più sereni, perché non saranno sottoposti al controllo di un altro funzionario, ma al controllo dell'autorità politica, fondamentale in un sistema democratico. L'elemento su cui insisto è che, alla fine, tutto risalirebbe all'autorità politica, proprio per far stare tranquilli.

Senatore Ramponi, questa riforma è stata concepita incentrandola su un punto chiave, cioè la responsabilità del Presidente del Consiglio.

lasciare al Presidente del Consiglio, come è accaduto nel passato, prima di questa legge, la possibilità di organizzarsi diversamente. Il punto è questo, sostanzialmente questo. Certo, se lei mi chiede se dal punto di vista operativo ciò sia necessario, francamente dico che è necessario, sì. Però, siccome per siccome per la prima volta la responsabilità non è più in capo ai Ministri vigilanti del passato (interno e difesa), ma viene tutta portata a livello del Presidente del Consiglio, a quest'ultimo, avendo tale aggravio di responsabilità,

riprendo il discorso del senatore Ramponi; Alleanza Nazionale in Commissione ha espresso l'orientamento che non c'è bisogno di avere un Ministro che faccia soltanto questo

niente? La figura del Sottosegretario, che non partecipa al Consiglio dei ministri, dà, a nostro giudizio, maggiore garanzia e vi è inoltre anche un maggiore impegno da parte del Sottosegretario che si occupa solo di questo.

a mantenere le deleghe; si tenga conto di questa nostra osservazione quando si sceglierà eventualmente un'autorità sotto il Presidente del Consiglio dei ministri.

farsi coadiuvare o di delegare queste funzioni ad un Ministro o ad un Sottosegretario. Non vi è un obbligo, ma una possibilità, una facoltà. Perché anche un Ministro? Perché già oggi è così, anche se il delegato dei Servizi non ha il rango di Ministro o non lo aveva con la seconda fase del Governo Berlusconi, però precedentemente vi sono stati Ministri che hanno ricoperto la carica di delegati ai Servizi di sicurezza. Ricordo il ministro Frattini e anche il ministro Mattarella, che era allora anche vice Presidente del Consiglio. Mi sembra quindi che il ventaglio di ipotesi viene rappresentato dal testo,

volevo precisare al relatore che è vero che già nella legge attuale non è specificato che il Presidente del Consiglio nomini e che, tuttavia, sono stati diversi i Ministri e i Sottosegretari incaricati, questo è verissimo, ma è altrettanto vero che, per esempio, il Presidente del COPACO, direi ormai per consuetudine, fa parte dell'opposizione.

Non c'è scritto che sono nell'ambito della Presidenza del Consiglio, non c'è scritto che sono dentro il Dipartimento di *intelligence* per la sicurezza; allora il mio suggerimento è di dare una veste organica, corretta e precisa a quello che voi avete già deciso costituisca nel complesso il sistema d'*intelligence*. Non lo volete fare? Pazienza, però a me pare con questo di non stravolgere proprio nulla. La posizione del mio Gruppo era di attenuare la

attenuarla perché ci sembra eccessivo che l'organo amministrativo - perché si tratta di un dipartimento della Presidenza del Consiglio - debba in qualche modo fare da tramite rispetto alle esigenze che i due Servizi operativi devono avere con il Governo e con il Presidente del Consiglio. La logica dei nostri emendamenti è in questa direzione: non si può dare potere assoluto al Dipartimento e quindi all'organo amministrativo di coordinamento e poi dare anche poteri di controllo, di spinta e addirittura un potere di "passacarte"

la prevalenza dell'organo di mezzo che, dovendo essere di coordinamento, deve consentire di più agli altri di avere contatto diretto con il Governo perché i veri

abbiamo redatto - e io ho sottoscritto come primo firmatario - una serie di emendamenti. Una parte di questi sono stati trasformati in un ordine del giorno; alcuni sono stati corretti e su altri, pochi, interverrò successivamente. I primi emendamenti in questione sono gli emendamenti 4.204, 4.208, 4.209 e 4.211 che vengono trasformati nell'ordine del giorno G4.100, relativo a un organismo molto importante e delicato istituito per la prima volta, per quanto mi risulta, all'interno della nostra storia costituzionale repubblicana. Si tratta dell'ufficio ispettivo e il timore è che possa essere creato un servizio segreto all'interno dei Servizi segreti. Quindi, si danno delle indicazioni, che sono state, per quanto mi risulta, accolte anche dal relatore, e che sottoponiamo anche al Governo, al fine di dare delle garanzie di autonomia ai membri di questo ufficio ispettivo, come indicato anche dal disegno di legge, anche a tutela nei confronti dei cittadini. In sintesi, si impegna il Governo, nell'adozione del regolamento relativo, a prevedere forme di selezione chiara e trasparente, che garantiscano capacità professionali e morali che tengano in considerazioni gli incarichi in precedenza svolti, in modo da evitare conflitti di interessi, contrasti istituzionali o rischi di copertura in fase di accertamento. Si impegna altresì il Governo a rendere noto al Parlamento il regolamento in questione e ad istituire appositi meccanismi a garanzia dell'indipendenza e autonomia di giudizio

qualora facesse esclusivo riferimento al decreto legislativo n. 286 del 1999. Chiedo pertanto l'attenzione del collega Saporito se è disponibile a trasformare tale emendamento in un ordine del giorno che inviti il Governo ad adottare per quanto compatibili, nell'attività di vigilanza del DIS sulle Agenzie, i criteri di cui al decreto legislativo n. 286 del 1999. Questo perché, signor Presidente, a nostro avviso richiamare espressamente le norme del citato decreto legislativo che concernono il riordino e il potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi

L'emendamento 4.206 punta a garantire trasparenza e correttezza nella gestione del personale dei Servizi, con la previsione di un consiglio per il personale ristretto, di emanazione mista del Governo e del Parlamento, che verifichi non le singole assunzioni o la collocazione di Tizio al posto di Caio all'interno del sistema dei Servizi, ma anche la correttezza dei sistemi di reclutamento e gestione del personale e quindi in qualche modo svolga una funzione di controllo inseribile in quella che già il Parlamento è chiamata a svolgere attraverso il Comitato parlamentare di controllo sui Servizi. Per questo, poiché risponde, lo ripeto, ad un'esigenza di oggettività anche nelle regole pur nella riservatezza del comparto, ne sollecito l'approvazione.

è un problema molto delicato. Noi abbiamo presentato questo emendamento perché a nostro giudizio, pur intendendo il Governo utilizzare la struttura del RIS a cui va il merito di avere, soprattutto all'estero, offerto un aiuto essenziale ai nostri Servizi e alle nostre Forze armate ed anche a tutti i cittadini, comunque per le missioni di pace, salvaguardandone anche la sicurezza fisica, ci è sembrato e ci sembra ancora molto riduttivo dire che il ruolo del RIS, e quindi le strutture, la rete all'estero, divenga semplicemente un fatto tecnico. Mi rendo conto che è stata fatta una riformulazione da parte del relatore e da parte del Governo che in qualche modo viene incontro a questa esigenza, però sarebbe bello se potessimo togliere la parola «tecnico» in modo da dare dignità al lavoro fatto in passato e soprattutto

non tanto al collega Saporito, che lo sa perfettamente, ma ai colleghi che non hanno partecipato ai lavori di Commissione, che nell'articolo 8, dove si parla appunto del RIS, la Commissione ha apportato una modifica piuttosto significativa proprio per andare al di là delle perplessità che il collega Saporito ha espresso qui e ha espresso già in Commissione. Credo che sia stato fatto un buon lavoro e quindi il testo dell'articolo 8 licenziato dalla Commissione merita di essere confermato nella sua integrità

che tale direzione sia costituita da rappresentanti dei Ministeri interessati ed esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori d'interesse: su questo posso anche essere d'accordo. Ma perché, perlomeno, non inserire anche esperti dell'attività di *intelligence*, cioè di quella struttura della quale la scuola fa parte? parte? Mi pare che l'emendamento 11.2, ancora una volta, non stravolga nulla, se è vera l'intenzione di prendere con serietà in considerazione le mie proposte e, nello stesso tempo, è estremamente opportuno, perché non vedo come si possa pensare di costituire una scuola, senza inserire nella sua direzione qualche rappresentante della struttura stessa per la quale la

uno soltanto perché fa riferimento all'attività della magistratura di acquisizione di documenti e atti. Il primo inserimento, la prima precisazione che chiedo e che chiediamo come Commissione giustizia nell'elaborare il parere fa riferimento al provvedimento del magistrato. Questi, quando chiede documenti, atti, cose oggetto della richiesta, non ha alcun altro obbligo: riteniamo invece più opportuno che l'autorità giudiziaria, proprio nell'ordine di esibizione, indichi i reati per i quali procede. Questo per evidenti motivi, ma soprattutto per il fatto che, se si dovesse trattare di reati per i quali non è opponibile il segreto di Stato, la particolarità dovrebbe risultare immediatamente all'esame di chi vede l'ordine di esibizione. Questa è la prima questione sulla quale mi permetterei di insistere, anche con i relatori. L'altra questione, riguardante la parte finale di questo articolo 15, con la sostituzione che propongo, concerne, ancora una volta, il comportamento della magistratura che chiede

«l'esame e la consegna immediata sono sospesi» con «l'esame» - in questo caso così generale - «è consentito, ma la consegna immediata è sospesa». Questo, da una parte, per facilitare le indagini, dall'altra, per rispettare il più possibile il segreto. In conclusione, ricordo che il magistrato è vincolato

di decidere. L'opzione che ha scelto la Commissione è che sia il Presidente del Consiglio, l'autorità politica ad avere nelle mani la capacità di decidere se il contenuto di un documento o di un atto debba essere conoscibile o meno,

è una cosa indispensabile, proprio per accertare se si tratti di un documento rilevante ai fini del processo e per valutare se debba chiedere, poi, l'autorizzazione al Presidente del Consiglio perché venga acquisito al processo medesimo. Bisogna dunque fare una netta distinzione tra l'esame del documento e l'acquisizione di quel documento al processo.

fiducia in un rappresentante delle istituzioni che sta svolgendo delle indagini per cercare di capire se ci sono dei reati in particolare commessi da qualcuno. Mi pare allora che le obiezioni che fa il relatore Sinisi in questo momento siano assolutamente al di là di ogni previsione e mettano in dubbio la correttezza del magistrato il quale, una volta esaminato il documento, potrebbe per sé quelle notizie fino a quando il Presidente del Consiglio non avesse sciolto la riserva sul segreto eccepito e non avesse deciso che quel documento può essere acquisito.

voglio dire due parole a sostegno di quanto ha sostenuto il relatore Sinisi. Il problema non è avere o no fiducia nel magistrato. La ragione per cui si appone il segreto non ha nulla a che vedere con la figura del magistrato, in quel momento non interessa minimamente. La ragione per la quale si appone il segreto o perché è opportuno che questi documenti non vengano letti da nessuno che non sia direttamente interessato alla condotta dell'operazione risiede

il magistrato, sul quale vi deve essere la massima fiducia, può leggere i documenti anche se non può utilizzarli: il ragionamento varrebbe anche nel momento in cui venisse apposto il segreto.

politico-parlamentare che, non siamo obbligati, ma cerchiamo di onorare anche in questa sede, per cui certe norme molto sensibili, secondo me, è opportuno che non vengano in ogni caso modificate, proprio perché

come dice giustamente il mio collega Polledri, allora cambiamogli la denominazione, chiamiamoli Servizi quasi segreti e andiamo avanti a discutere, perché o ci sono o non ci sono, o si ritiene che ad uno Stato, per quanto democratico, occidentale, con rappresentanza parlamentare, eccetera,

queste situazioni intermedie per controllare i Servizi in qualche modo, ma semplicemente facciamo una bella discussione parlamentare, decidiamo che non servono più, li togliamo e fine della trasmissione, c'è la polizia ordinaria che segue le cose normalmente; poi, quando ci sono problemi particolari, diremo agli alleati, agli altri Paesi che non siamo d'accordo con loro, che le cose segrete non le facciamo, trattiamo tutti alla stessa maniera con la giustizia ordinaria, con le forze dell'ordine ordinarie e fine della trasmissione. Se invece riteniamo che i Servizi segreti debbano esserci per mille ragioni, mille ragioni, sono convinto che ognuno di noi, anche chi è completamente d'accordo con la loro esistenza, avrebbe comunque tutta una serie di eccezioni, di cose da proporre, eccetera, però ci sono delle questioni che ad un certo punto o si accettano o non si accettano. Mi pare che alla fine comunque il Presidente del Consiglio - lasciando perdere

che non ci convincono completamente dal punto di vista della trasparenza democratica, alla fine c'è quest'uomo, o questa donna, che in qualche modo fa da garanzia finale. In questo senso, come dire, una sorta di aggiustamento accettabile il fatto che un Paese, che pur deve garantire tutta una serie di princìpi logici, ovvi, assolutamente non discutibili, abbia un un organismo che in qualche modo si comporta in maniera un pochino particolare e però alla fine ha comunque un qualcuno che verifica e garantisce per l'istituto stesso. Detto questo, vorrei veramente che in quest'Aula si smettesse di santificare la magistratura. Non è che in Italia ci sono 59 milioni di persone normali e poi 10.000 persone *super partes* in odore di santità, che appena defunte vengono immediatamente beatificate e iniziano l'*iter* per la santificazione. Il magistrato è un uomo come un altro: che faccia il suo mestiere e basta! Ogni volta in quest'Aula ci si alza a dire «questi servitori della patria»: perché, gli altri non sono servitori della patria e dello Stato? Tutti gli altri che sono dipendenti pubblici e non sono magistrati non sono servitori dello Stato? I muratori che vanno sui ponteggi tutti i giorni non sono servitori dello Stato? Tutti quelli che pagano le tasse non sono servitori dello Stato? *(Applausi dal Gruppo* *LNP)*. Smettiamo di raccontare la storia che c'è una categoria di persone che

dicendo ad un marocchino che quando in Italia si sale sul tram si paga il biglietto, ma il marocchino evidentemente non lo sapeva. Detto ciò, se al magistrato Forleo andasse in mano un fascicolo che per la maggior parte dei magistrati normali

che hanno studiato come altri, magari anche meno di tanti altri, che hanno vinto un concorso (credo in gran parte in maniera regolare, in parte minoritaria forse non così regolare), che esercitano un mestiere come un altro,

che in automatico hanno diritto di vita o di morte su tutto e possono fare quello che vogliono è una cosa, questa sì, che in un Paese democratico non esiste assolutamente. Entrando poi nel merito della questione, mi sento a questo punto più garantito da un funzionario dei Servizi segreti che alla fine è comunque controllato dal Primo ministro che fa ciò che ritiene giusto fare, piuttosto che avere una serie di pazzi che possono avere accesso a qualunque cosa e mettere in pericolo, com'è stato fatto qualche mese fa,

15.201, io sono di "manica larga" sugli ordini del giorno, ma credo che in questo caso la trasformazione in ordine del giorno francamente non sia possibile, perché la richiesta è estremamente chiara, o è bianco o è nero. Si tratta di compiere una scelta o con riferimento alla politica o con riferimento

Signor Presidente, ho ascoltato con molto interesse le argomentazioni del collega Casson e devo dire che, dal punto di vista della necessità che la giustizia possa utilizzare, ai

Il problema, a mio modo di vedere, è quello di stabilire lafunzione del segreto di Stato, che non è il segreto di un Governo,

mi trovo in linea con quanto affermato dal relatore, perché egli ha operato la scelta di una prevalenza di un interesse generale che può essere messo in pericolo non perché vi siano dei disonesti, ma perché il fatto stesso della conoscenza

degne di considerazione. Credo che l'interesse superiore dello Stato, e non di un Governo, che copre con il segreto una realtà che lo riguarda all'interno e all'esterno, nelle sue relazioni internazionali,

così come è stata predisposta all'interno della Commissione competente e per tenere fede all'accordo di procedere su questa strada. Quindi, le considerazioni svolte dal senatore Biondi

recita: «Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in

modo, non capisco perché alcuni giornalisti non possano essere oggetto anche loro di un'azione da parte dei Servizi che - voglio ricordarlo - agiscono per la tutela e l'interesse dello Stato. Mentre per la parte politica, che è elettiva, posso ancora capirlo, per queste altre due categorie non riscontro una specialità nel loro essere che consenta addirittura di essere al di fuori di iniziative mosse per la tutela delle istituzioni e la difesa della società.

Presidente, a mio parere esiste un'incongruità formale e sostanziale nel comma 5. Praticamente, in esso le condotte previste al comma 1 sono vietate nei luoghi dove si svolgono determinate funzioni.

dal quale sono emerse sensibilità, esigenze, rappresentazioni diverse, spesso convergenti, altre volte divergenti, su questi temi. Evidentemente,

di rappresentare e di regolamentare un'esigenza che in altri Paesi è già regolamentata. Però, esistono dei precisi binari. Come dicevo, è chiaro che su ogni parola ed espressione possono

calibratura, sulla quale non necessariamente dobbiamo essere d'accordo, ma che rappresenta nel campo delle scelte politiche un risultato di sostanziale equilibrio.

ho ascoltato con attenzione i relatori. Non si tratta di concedersi qualcosa reciprocamente, ma di capire se questo snodo consentirà ai Servizi, in un quadro di garanzie democratiche, di funzionare in modo adeguato. Avevo presentato, poi ritirandolo, un emendamento interamente soppressivo del comma 5. 5. Il comma 2 fissa dei limiti molto rigorosi, in termini di garanzie funzionali, considerando sempre illecite determinate condotte che sono descritte La cronaca recente e meno recente ci informa di collusioni e complicità nei confronti di attività terroristica anche in alcune sedi di organizzazioni sindacali. Mi chiedo perché si debbano legare le mani ai Servizi e impedire loro di acquisire informazioni, per esempio, in questi luoghi o realtà che hanno manifestato tali elementi di preoccupazione. Si vuol mantenere in piedi il comma 5? Come ho già detto, proprio in un'ottica di condivisione massima del testo, ho ritirato l'emendamento soppressivo del comma 5, ma almeno si permetta in casi eccezionali, così come prevede l'emendamento 17.8 a mia firma, che il Presidente del Consiglio si assuma la responsabilità di autorizzare lui, lui, senza dare questa discrezionalità al direttore del Servizio, la possibilità di acquisire informazioni in queste sedi. Tra queste sedi ho escluso, ovviamente, il Parlamento e le sedi rappresentative del territorio, ma ho lasciato le sedi di partiti politici, di organizzazioni sindacali o di giornalisti. Questo perché, ripeto, spiace ricordarlo, ma i fatti che hanno descritto episodi criminali terroristici negli ultimi tempi non rassicurano da questo punto di vista. Per questo motivo sostengo la necessità di approvare l'emendamento

è veramente un appesantimento di procedura di cui non vi è nessuna ragione sostanziale; vi è già una procedura autorizzativa che ha una sua compiutezza nei commi precedenti, non riesco a capire per quale motivo al Presidente del Consiglio vada chiesto se è proprio sicuro.

proposti) è molto rilevante perché, pur prevedendo una serie di regole che verranno attuate in via regolamentare, tuttavia si riferisce al personale dei Servizi di informazione per la sicurezza, cioè alle agenzie e al DIS. Tale articolo è importante proprio perché definisce una nuova cultura dell'*intelligence*, soprattutto quella cultura del limite che - vorrei sottolinearlo - qualcuno mi sembra non abbia ancora colto. Essa si riferisce al limite dato dai princìpi costituzionali e dalle normative vigenti; quindi, non c'è nessun Presidente del consiglio che ha diritto di vita e di morte.

il trattamento economico degli operatori di sicurezza. È importante, a mio avviso, perché mantiene all'interno dei Servizi di informazione per la sicurezza

e, comunque, non un'attrattiva dei Servizi di informazione e sicurezza nei confronti di dirigenti o qualifiche alte delle forze dell'ordine o delle Forze armate o, comunque, di personalità anche esterne al mondo militare o di Queste motivazioni ci hanno spinto a sostenere la necessità di tutelare l'attuale trattamento economico, quello esistente all'interno delle risorse finanziarie già previste dalla dalla normativa vigente. Credo che l'articolo abbia una particolare rilevanza perché se è vero che i fatti recenti hanno creato un senso di sfiducia e di sospetto nei confronti degli operatori di sicurezza, è altrettanto vero che questo clima deve cambiare all'interno stesso delle strutture; se non si prevedono infatti, anche in via regolamentare norme di trasparenza e minore discrezionalità, quindi minore soggettività, non c'è neanche una democrazia vera all'interno degli degli stessi Servizi. Ciò crea situazioni patologiche che hanno riflessi altrettanto devianti e patologici nelle situazioni di rapporto con l'esterno. Si tratta di un punto estremamente rilevante dell'articolo 21 perché, secondo me, sono state definite norme più trasparenti e più chiare che consentono anche di dare fiducia a quegli operatori che la meritano; le responsabilità devono essere punite, ma è altrettanto vero che gli operatori di sicurezza leali nei confronti dello Stato e dell'interesse nazionale vanno garantiti.

all'interno di quest'Aula una difesa comune; da qui il motivo per cui l'emendamento appena illustrato dalla senatrice Villecco Calipari è sottoscritto anche da me.

Non sfugge a nessuno che all'interno di quest'Aula è stato trovato un fronte comune, che speriamo possa raccogliere il consenso anche del Governo su un aspetto delicato come quello del trattamento economico relativo al personale impiegato nei Servizi di sicurezza. Noi crediamo che, nell'ottica del condiviso impegno internazionale che vede il nostro Paese in prima linea nella lotta al terrorismo, la proposta riforma del comparto *intelligence* dovrebbe tendere a migliorare e a rendere più efficiente le varie articolazioni dei nostri Servizi di sicurezza. È universalmente riconosciuto che la delicatezza dell'attività svolta dagli appartenenti ai Servizi e i rischi che essa comporta giustificano un trattamento economico differenziato. Tenuto conto che l'attuale retribuzione per la grande maggioranza del personale, considerate tutte le voci che la compongono, è superiore di quel tanto che crea quel minimo, forse giusto, incentivo per il personale meritevole ad intraprendere una nuova carriera, ma che spesso al rientro nell'amministrazione di provenienza comporta anche disagi e svantaggi per chi ha svolto l'attività d'*intelligence*, noi ci domandiamo perché mai un lavoro così difficile, spesso pericoloso, silenzioso e senza nessuna tutela il più delle volte debba essere svolto senza quel giusto premio a chi mette a repentaglio non solo la propria sicurezza personale, ma spesso l'equilibrio della propria vita, di quella familiare e delle tante cose che noi forse nemmeno conosciamo, che vengono sacrificate dagli appartenenti ai Servizi sull'altare dell'interesse nazionale e dell'attività particolarmente meritevole che da loro viene svolta. Se allineare le retribuzioni del comparto *intelligence* a quelle delle forze di polizia sottintende un intento punitivo per il primo in virtù di un accettabile pregiudizio ideologico, ravvivato ahimè da recenti avvenimenti di cronaca, è invece corretto rendersi conto che non si può oggettivamente pretendere, in un momento così delicato, un rinnovato impegno professionale da parte di chi si vorrebbe ridimensionare sotto l'aspetto economico. Ho una certezza: se il nostro Paese é stato risparmiato in questi anni da fatti di cronaca legati al terrorismo internazionale che hanno attentato alla sicurezza di altri Paesi, che come noi sono impegnati allo stesso modo sullo scenario internazionale, questo è dovuto alla grande capacità e al grande merito di tanti uomini e molte donne che hanno lavorato con grande competenza e che hanno risparmiato al nostro Paese sangue e dolore che, invece, ad altri Paesi non è stato risparmiato. Penso anche che all'interno di questa nostra discussione così equilibrata e condivisa, per la volontà di entrambe le parti che oggi si confrontano su questo delicato tema,

dovrebbe ringraziare le persone, uomini e donne, che lavorano per la nostra sicurezza nell'ottica di un impegno quotidiano che non viene mai meno e che noi non premiamo abbastanza. In tutti i settori informativi dei Paesi occidentali la componente *humint* (la *human* *intelligence*, cioè l'intelligenza umana che fino all'11 settembre aveva riscontrato un malaugurato calo di interesse e di investimenti a vantaggio della tecnologia più avanzata) sta riottenendo il posto di preminenza che merita, in quanto rappresenta una delle componenti più utili nelle attuali azioni di contrasto alle minacce

mortificherebbe la professionalità e la motivazione nella stragrande maggioranza degli operatori dell'*intelligence* italiana. Non possiamo, allora, andare in controtendenza rispetto

di ragionare nuovamente sull'utilizzo delle risorse economiche, premiando quelle legate all'intelligenza e al merito e alla capacità dei nostri appartenenti. Infine, se le esigenze di bilancio impongono l'invarianza degli oneri a carico dell'erario per l'attuazione di questa riforma, è pur vero che molti comparti dei nuovi organismi informativi sono stati ridisegnati proprio con l'intento di ottimizzare l'impiego dei fondi e di ridurre costose sovrapposizioni dei ruoli. Il nostro sforzo, quindi, dovrà essere concentrato ad evitare che le innovazioni previste nella nuova riforma sui Servizi, in virtù dell'invocata mancanza di risorse, vengano letteralmente addebitate a quella maggioritaria aliquota di personale che svolge le proprie delicate funzioni con abnegazione e senso del dovere, assicurando al Paese una credibile cornice di sicurezza. Presidente, o noi crediamo nel valore della nostra *intelligence* rispetto alla sicurezza del nostro Paese oppure non ci crediamo. Se ci crediamo dobbiamo dare merito, riconoscenza e fiducia a quegli uomini che finora, comportandosi correttamente nel rispetto della legge, hanno garantito al nostro Paese un po' di sicurezza in più.

al quadro generale dei Servizi e all'organizzazione dell'*intelligence*, relativamente all'articolo 21 abbiamo detto in maniera chiara (lo hanno ripetuto tutti i colleghi di Alleanza Nazionale che sono intervenuti) che il problema del personale diviene centrale in questo disegno di legge, anche per la clausola dell'invarianza della spesa. Abbiamo quindi tentato di affrontare

e ci eravamo riservati una formulazione diversa. La stessa collega Villecco Calipari aveva promesso di tentare di risolvere questo problema.

fanno i colleghi al regolamento generale, che tratterà compiutamente questa materia, ci sentiamo soddisfatti e ritiriamo

l'espressione «nemmeno saltuariamente». Questo inserimento non è assolutamente un attacco né uno stravolgimento dell'attività dei Servizi, anzi è una formulazione letterale

Dico questo con riferimento ai membri del Parlamento ma in particolare ai magistrati, perché ritengo assurdo che un magistrato possa diventare fonte o talpa dei servizi di sicurezza e questo proprio a garanzia proprio della terzietà e dell'indipendenza. Sono convinto che nessuno di noi, e nessun cittadino, potrebbe credere nella terzietà e indipendenza di un magistrato che sia fonte o talpa dei Servizi di sicurezza. Quindi, al di là

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho una riserva di fondo sull'impostazione di questa riforma e in sede di voto finale la appaleserò. Anche per questo mi sono finora astenuto dall'intervenire su singoli aspetti. Prendo la parola, però, sulla questione sollevata dalle colleghe Villecco Calipari e Bonfrisco perché la considero di importanza decisiva. In questi anni di pratica esperienza nella lotta al terrorismo internazionale e alla criminalità organizzata, noi abbiamo visto emergere come non mai la preminenza del fattore umano e della intelligenza umana proprio nel momento in cui le tecnologie più sofisticate raggiungevano limiti fino a poco tempo fa impensabili. La verità è che sistemi di sicurezza anche tecnologicamente carenti funzionano bene se possono disporre di intelligenza umana e fattore umano ben motivati. Al contrario, le le strutture tecnologicamente più avanzate si rivelano inefficaci in carenza di un fattore umano motivato. Allora su questo punto bisogna insistere guardando innanzi tutto alle modalità di reclutamento del personale ma, con pari attenzione, alle modalità di formazione e di retribuzione dello stesso.

non era qualificato dal punto di vista professionale ma tendeva soltanto a ottenere determinati livelli retributivi. Ora, nel momento in cui noi, con questo disegno di legge, poniamo la questione di una grande professionalità e qualificazione degli addetti ai Servizi, è chiaro che dobbiamo considerare fondamentale anche il trattamento economico perché, come giustamente ha sostenuto l'*ex* ministro Pisanu, in questa fase il ruolo degli addetti ai Servizi e il loro profilo professionale e morale, la loro capacità di coinvolgimento nell'attività che svolgono è fondamentale. anche le recenti esperienze, soprattutto dopo l'11 settembre, hanno dimostrato che le tecnologie svolgono sì un ruolo di grande importanza, ma poi occorre l'uomo in carne ed ossa che sul teatro d'azione e d'intervento risponda a determinati requisiti. Ecco perché non possiamo, nella maniera più assoluta, far sì che far sì che ci sia un processo di appiattimento per quanto riguarda lo *status* del personale del personale dei Servizi sotto l'aspetto economico. Ecco perché, a mio avviso, l'emendamento senatrice Villecco Calipari, pongono una questione molto seria a cui successivamente non ci si potrà sottrarre in fase di regolamento.

Innanzitutto, signor Presidente, se mi consente vorrei sottolineare il fatto che sono orgoglioso di vivere in un Paese nel quale la Marina militare, la Guardia costiera e tutti coloro che sono in mare si diano da fare e si impegnino per salvare vite umane quando ciò è necessario.

a queste norme che finalmente mettono ordine nel reclutamento del personale, stabilendo princìpi e criteri cui dovrà uniformarsi

Ho ascoltato con attenzione l'intervento del collega ed ex ministro dell'interno Pisanu. Ho colto un elemento di critica nei confronti dell'impianto complessivo della legge che so riferibile alla scelta che si è compiuta in questo testo di legge di mantenere comunque separate due strutture che possano concorrere assieme all'attività di informazione per la sicurezza. Vorrei invitare il collega Pisanu a considerare che questo è un punto di mediazione tra posizioni che erano in partenza diverse

Per questo motivo, confido che, sulla base della considerazione dei punti di partenza di ciascuno e della mediazione che qui si è operata, anche il collega Pisanu voglia assicurare il suo voto favorevole a questo testo.

«invita il Governo ad indicare nei regolamenti la percentuale massima dei soggetti da assumere per chiamata diretta». Abbiamo ritenuto di non dover portare nella legge le percentuali, ma di affidare questo compito ai regolamenti, lavoro che abbiamo svolto in Commissione. Coerentemente, ritengo sufficiente un ordine del giorno che inviti il Governo ad indicare nei regolamenti il numero massimo di soggetti da assumere per chiamata diretta.

e che è bene non indicare nella legge la percentuale di coloro che vanno assunti per chiamata diretta; ma l'emendamento non indica tali percentuali, bensì demanda ai regolamenti di stabilire l'aliquota di personale che deve essere assunto in termini massimi per chiamata diretta. L'ordine del giorno andrebbe nella stessa direzione, per cui non vedo perché non si debba scrivere già nella legge.

Se c'è una cosa che, quanto a gestione del personale, ha sollevato perplessità negli ultimi tempi a proposito dei Servizi è proprio una certa discrezionalità - usiamo un eufemismo - nella chiamata diretta.

perché il precedente, che è stato respinto, indicava invece una quota fissa. Ora continuo a non capire perché quello che dovrebbe essere contenuto nell'ordine del giorno non possa già stare nell'emendamento.

il sostegno e la firma dei colleghi Saporito e Mantovano. Mi sembra di aver capito che anche i colleghi di Forza Italia stiano ritirando il loro emendamento.

ci sono tre sentenze della Corte costituzionale (la n. 110 del 1998, la n. 410 del 1998 e la n. 287 del 2000) che fanno divieto all'autorità giudiziaria di utilizzare informazioni e notizie non consentite e coperte da segreto direttamente o indirettamente. Quindi, c'è una pacifica giurisprudenza della Corte costituzionale che afferma che l'autorità giudiziaria non possa svolgere

Signor Presidente, la giurisprudenza e anche la dottrina sono solo parzialmente conformi. Comunque, per le motivazioni che ho espresso prima, ritiro l'emendamento

più opportuno un numero inferiore di componenti del Comitato per tutelare meglio le esigenze sia di speditezza dei suoi lavori, sia di riservatezza, requisito fondamentale degli stessi.

insisto sull'emendamento 31.208 rispetto al quale vorrei conoscere

Mi ricollego alle osservazioni svolte in sede di discussione generale e credo sia utile all'equilibrio complessivo del provvedimento che i poteri del Comitato parlamentare di controllo siano rafforzati, così come risulta da questa norma, poiché ciò costituisce un sistema di contrappesi e di bilanciamento: da un lato, introduciamo norme che danno maggiore efficienza all'attività dei Servizi fino alle cosiddette garanzie funzionali e, dall'altro, rendiamo più penetrante il potere di controllo del Comitato parlamentare.

questa parte concerne i poteri del Comitato parlamentare di controllo, che potrà quindi anche sentire gli appartenenti all'ufficio ispettivo, di cui si è parlato all'inizio della seduta odierna; inoltre, le persone ascoltate dal Comitato parlamentare di controllo

Presidente, sono un po' sorpreso della circostanza che, a fronte di una disponibilità a trattare la materia

Tale Comitato, però, non può basare la sua attività sulla buona volontà di coloro che di volta in volta vengono ascoltati. La buona volontà si può anche presumere;

il comportamento sleale nei confronti del Parlamento nel suo insieme, che in quel momento è rappresentato dal Comitato dei Servizi, si trova privo di qualsiasi sanzione. Immagino quale possa essere l'obiezione, perché è stata già in qualche misura formulata nella discussione in Commissione: si afferma che prevedere una sanzione, cioè il richiamo agli articoli dal 366 al 384-*bis* del codice penale, significa in qualche misura riconoscere al Comitato parlamentare di controllo poteri simili a quelli delle Commissioni parlamentari di inchiesta, che hanno necessità, per dettato costituzionale, di un'apposita legge istitutiva. Non è necessariamente questa la conclusione. Infatti, quando un soggetto, che non ha una veste di indagato o di indagabile in sede processuale, viene chiamato a riferire fatti di cui si presume sia a conoscenza al Parlamento, il sacrosanto rispetto nei confronti del Parlamento che esercita la funzione di controllo che gli è riconosciuta dalla Costituzione e dalla legge gli impone di dire il vero; se non dice il vero, la cosa non può rimanere senza effetto. Da ciò, il richiamo di queste disposizioni, che non sono soltanto quelle della falsa testimonianza, ma anche quelle che nel giudizio consentono, a chi si trovi in condizioni particolari, ad esempio perché parente di un soggetto potenzialmente leso da una sua dichiarazione, di esimersi dal riferire ciò di cui è a conoscenza. Trovo squilibrato un parere contrario a questa norma, che priverebbe il Comitato di controllo

Presidente, non essendo personalmente sospettabile di una convergenza con il collega Mantovano dettata da ragioni politiche estrinseche rispetto al merito della specifica questione trattata,

da parti politiche diverse, di un rafforzamento dei poteri del Comitato parlamentare di controllo. Fermi restando lo spirito di mediazione e la necessità di trovare un punto d'intesa, se queste considerazioni potessero essere oggetto di esame e rivalutazione da parte

sottendenti all'emendamento sono apparse, e sono ancora, del tutto infondate. La questione ha un profilo di costituzionalità,

una previsione specifica, all'articolo 82, in base alla quale soggetti rappresentativi del Parlamento

dichiarare che è necessario avere grande considerazione del personale; qualcuno l'ha chiamato «la componente *humint*», qualcuno «l'intelligenza della struttura» e non v'è dubbio che, in realtà, la componente umana è sempre la più delicata in tutte le organizzazioni.

Seconda considerazione: siamo in una Repubblica che istituzionalmente si dichiara Repubblica parlamentare. Ho udito accenti favorevoli nei confronti delle norme di legge che prevedono un'intensificazione, una maggiore incisività

Detto questo, allora, se è vero che la persona ha un'importanza fondamentale, se è vero che è estremamente opportuno che il Parlamento possa recitare questa sua funzione come si deve,

e dei direttori e dei vice direttori dei Servizi di sicurezza. In questo Paese capitano cose veramente strane. Come ho già ricordato, siamo una Repubblica parlamentare dove il Parlamento recita la sua funzione fondamentale, ma, per esempio,

Paesi di alta importanza e, comunque, di un rappresentante dello Stato italiano, oppure quella del Capo di stato maggiore della Difesa, o dei diversi Capi di stato maggiore, mentre poi il Parlamento si esprime

da protagonista, di controllo e anche - direi - di dovuta assunzione di responsabilità, riconosciamogli la facoltà di esprimere un suo parere sulle scelte del Governo per incarichi davvero importanti e cominciamo da questa volta.

normativo vuole che il Comitato parlamentare nella sua interezza abbia un potere di denunciare all'autorità giudiziaria per fatti costituenti reato. Credo che, così come è scritto, sottragga questo potere di denuncia ai singoli membri del Comitato. A mio avviso, il pubblico ufficiale in quanto tale può, anzi deve, fare denuncia dei reati di cui è a conoscenza; per questo lo invito al ritiro perché addirittura mi sembra contrario agli stessi propositi che egli stesso intendeva prefigurarsi.

si tratta di una questione molto delicata ed è quella che riguarda una formulazione dell'articolo 202 del codice di procedura penale. Ha attinenza all'obbligo per i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. di Stato. Anche recenti vicende di cronaca giudiziaria ci hanno dato contezza di come in certe situazioni il diritto alla difesa di una persona indagata o imputata (diritto garantito dall'articolo 24 della Costituzione) cozzi in maniera fortissima con l'obbligo di questa norma del codice di procedura penale. Propongo questa modifica non soltanto a livello personale, ma perché ne abbiamo discusso ampiamente in sede di Commissione giustizia redigendo anche un parere in tale senso e ritenendo che il diritto alla difesa sia un diritto di qualsiasi persona tutelato in maniera amplissima che non può essere assolutamente compresso. Anche in situazioni di questo tipo, quindi, bisogna dare la possibilità alla persona imputata di un reato di difendersi e di scegliere se dichiarare o meno senza possibilità di incorrere in sanzioni di qualsiasi tipo: penale, amministrativo, disciplinare o di altro genere. Credo, quindi, che in nome dell'affermazione del diritto alla difesa costituzionalmente garantito

Questa larghissima dottrina dice che lo *ius* *tacendi*, cioè il diritto dell'imputato e dell'indagato ad avvalersi della facoltà di non rispondere, copre interamente la possibilità che siano addotte motivazioni di tipo diverso rispetto a questa facoltà che gli viene garantita dall'ordinamento. Per questo questa dottrina appunto dice che il segreto di Stato può essere o non essere argomentato come motivazione dello *ius* *tacendi*, fermo restando che è del tutto ininfluente e indifferente. Voglio soltanto aggiungere che il fatto che c'è un riferimento al solo testimone nell'articolo 202 del codice di procedura penale, con riferimento al segreto di Stato, dovrebbe far riflettere anche i presentatori perché il segreto di Stato, sotto questo profilo, non è l'unico caso che disciplina appunto la prerogativa del testimone e non dell'imputato o dell'indagato. Noi andremmo a creare un sistema diverso per il segreto di Stato rispetto a quello previsto per il segreto professionale e d'ufficio. Non si può modificare soltanto l'articolo 202 del codice di procedura penale senza modificare analogamente gli articoli 201 e 200 e tutti gli altri articoli che fanno riferimento al segreto che, come ho detto, riguardano solo il testimone. Presidente, per queste ragioni credo che la norma, laddove introducessimo una questione di questa natura, cioè che l'imputato o l'indagato non possa addurre il segreto di Stato come motivazione o debba essere superato rispetto alla motivazione che egli porta per avvalersi o meno della facoltà di non rispondere, è una limitazione che genera confusione nel sistema. Non può essere riferita solo al segreto di Stato e, peraltro, come ho detto, secondo una larghissima

tra l'altro, anche nella giurisprudenza e nella dottrina i pareri sono discordi. Ritengo comunque di dover privilegiare il diritto alla difesa costituzionalmente garantito e quindi per quanto mi riguarda mantengo questo emendamento.

di tutti i documenti classificati che concernono gli ordini impartiti dall'Esecutivo ai Servizi e le spese sostenute. Quindi, invito il Governo a documentare questa attività in maniera chiara ed efficiente. Se il collega Vitali accetta la trasformazione del primo periodo del secondo comma in ordine del giorno il parere sarebbe favorevole.

sui temi del segreto di Stato che è stata effettuata da un gruppo di giuristi attivati dall'Associazione familiari delle vittime del 2 agosto. Com'è noto a questa Aula, anche nelle legislature precedenti tale associazione aveva proposto l'abolizione del segreto di Stato per i reati di strage.

L'emendamento 42.0.200 sottopone al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica tutti gli accordi internazionali segreti o riservati. È una materia molto complessa, molto delicata e nuova rispetto al testo che abbiamo discusso fino ad

che le norme che vengono introdotte relativamente all'acquisizione di atti coperti da segreto di Stato e le relative limitazioni si applicano, così dice l'emendamento, alle acquisizioni probatorie successive all'entrata in vigore della presente legge. Dovrebbe essere pacifico perché vige il principio processuale del *tempus regit actum*, peraltro, siccome in precedenti leggi è successo che sono state date ed effettuate valutazioni diverse, credo che sia opportuno per la migliore comprensione e applicazione di tutti l'adozione di questo emendamento.

Signor Presidente, colleghi, questa riforma giunge al voto finale dopo un cammino piuttosto lungo e dopo lavori serrati in Commissione. Si tratta di una riforma organica che vede la luce dopo parecchi decenni da quella del 1977. Non esitiamo ad affermare che il lavoro svolto è stato lungo e faticoso e ha prodotto modifiche anche sostanziali rispetto alle proposte iniziali. Esso mostra nel suo impianto le novità dell'individuazione di un centro politico unico di responsabilità nel Presidente del Consiglio. Avremmo voluto ulteriormente migliorare il testo, anche relativamente a questo aspetto, attraverso gli emendamenti presentati in Aula. Tuttavia, siamo sufficientemente soddisfatti del risultato finale. Si tratta di una riforma che non può guardare al contingente, all'attività processuale, ma si rivolge ai decenni successivi del Paese, per regolare uno degli aspetti più delicati di uno Stato democratico, ossia il controllo, la responsabilità, l'efficacia e l'efficienza dei Servizi Purtroppo, - vogliamo dirlo ancora una volta e non è un accusa che tende ad una criminalizzazione dei nostri apparati - la storia di questa giovane Repubblica spesso contrassegnata non da Servizi affidabili o attaccati alle istituzioni democratiche, ma da gravissime deviazioni dei Servizi stessi a partire dal dopoguerra sino ad oggi. Come dicevo prima, apprezziamo l'impianto della riforma e siamo soddisfatti per avere ottenuto alcuni risultati nell'interesse generale, non di una maggioranza

anche se riteniamo che si sarebbe potuto maggiormente rafforzare l'impronta del provvedimento, soprattutto - lo ripeto - per quanto concerne il ruolo del Presidente del Consiglio e le sue prerogative che intendiamo debbano essere irrobustite (compresi i margini entro i quali egli assume le sue determinazioni con nettezza), ribadiamo il giudizio complessivamente positivo rispetto ai lavori di quest'Aula e agli sforzi messi in atto per realizzare una riforma di cui si sentiva fortemente l'esigenza e sulla quale il nostro Gruppo voterà convintamente a favore.

Signor Presidente, rivolgo innanzitutto un ringraziamento ai relatori per il lavoro che hanno svolto e che, riepilogato, ha sostenuto il lavoro di convergenza anche dei componenti della Commissione. Tuttavia, il voto favorevole che sto annunciando non ignora alcune ragioni critiche che andrò molto sollecitamente Il testo esitato dal Senato, dopo quello della Camera, è il punto di incontro di esigenze diverse, a volte contrapposte e contraddittorie. Permangono due concezioni antitetiche nell'affrontare un argomento delicato e complesso qual è quello dell'organizzazione dei Servizi. Vorrei ricordare che la riforma del 1977 fu il risultato non di un compromesso (è una parola che è diventata molto dispregiativa; anzi viene talvolta usata in termini accusatori), ma di onorevole compromesso tra l'allora ministro dell'interno Cossiga e il ministro dell'interno «ombra» del Partito Comunista Pecchioli. Eravamo alla vigilia di una grande svolta politica, quella compiuta dal Partito Comunista che accettava l'integrazione e l'inserimento nella pienezza del sistema democratico (con le sue regole) e che, soprattutto, aveva accettato, con una proclamazione ufficiale in Parlamento, l'adesione alla NATO che era stata un argomento di grande contestazione e contrasto tra le forze democratiche, i partiti di centro, lo stesso Partito Socialista e il Partito Comunista nei lontani anni Quaranta Nel 1977, c'è una svolta politica e, quindi, si può affrontare il problema della riorganizzazione dei Servizi in una chiave nuova: vi è un partito che ha rappresentato, con la propria adesione al sistema comunista e al blocco sovietico, un punto interrogativo; quel punto interrogativo non si pone più e insieme si lavora,

la modifica introdotta non parla più della sicurezza democratica all'interno del Paese, ma della sicurezza della Repubblica. Quest'ultima, però pone un valore sul quale pende sul quale pende un punto interrogativo: oggi la riorganizzazione dei Servizi tiene conto di un mutato equilibrio internazionale. È caduta la cortina di ferro e non vi è più un nemico dal quale guardarsi in Europa (e non vi dovrebbero essere più nemici); abbiamo sperato tutti che fosse finita la storia con il titolo di Furet, ma sappiamo che non è così e vi sono altri problemi, come il terrorismo. Di fronte a quest'ultimo problema, che per di più ha la connotazione islamica, è ovvio che la ristrutturazione dei Servizi debba anche superare

adesso è stato approvato un emendamento presentato dal senatore Brutti, che ha rafforzato ulteriormente i poteri del Comitato parlamentare di controllo. Mi sorge una domanda: ma è compatibile

lo Stato democratico - quale si va costruendo, non soltanto qual è stato costruito, sulla separazione dei poteri - poi abbia un punto culminante, che è la toga? Non sono un uomo che ha mai fatto polemiche sulla magistratura, anzi, ho un altro servizio nella mia vita politica; questa, però, è una contraddizione che, in prospettiva, stabilirà un punto interrogativo molto serio

delicatissimo, intorno al quale non sono mancate, anche di recente, polemiche

in cui si confrontano la necessità della riservatezza, da un lato, e l'esigenza della trasparenza e dell'informazione nei confronti dell'opinione pubblica, dall'altro. Certamente, questo è un tema importante nel mondo di oggi, non meno che in quello di ieri: in qualche intervento che mi ha preceduto, si ricordava, appunto il mondo della guerra fredda, diviso in due blocchi. sicuramente la situazione è diversa, ma in ogni caso anche nel mondo di oggi non vi è dubbio che un grande Paese abbia bisogno di apparati di sicurezza efficienti, perché un apparato di sicurezza in in grado di svolgere con efficacia il proprio ruolo è certamente uno snodo fondamentale nella tutela dello Stato democratico. Noi esprimiamo un giudizio complessivamente positivo su questo testo, che ha cercato di affrontare le questioni con equilibrio - ed io credo sia apprezzabile il lavoro svolto in Commissione ed anche, per così dire, la convergenza che su questo testo si è potuta verificare tra

accettabile e, ripeto, positivo. Notiamo che sono stati affrontati con attenzione e io penso con risultati accettabili accettabili i passaggi più delicati di questa problematica: rilevo in particolare, per esempio, tutta la parte relativa all'identità di copertura, alle attività simulate, di cui agli articoli 24 e 25, al trattamento delle notizie personali di cui all'articolo 26, alla tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari, alle comunicazioni di servizio e al delicatissimo problema quindi del segreto di Stato, che viene affrontato nell'articolo 28. Su qualche punto Su qualche punto forse avremmo preferito soluzioni non del tutto coincidenti, ci sembra senza dubbio che il risultato si possa nel complesso accettare. Così pure sottolineiamo il Capo IV, sul controllo parlamentare, che, come è chiaro a tutti, è il passaggio che dà equilibrio al sistema, perché accanto all'apparato di sicurezza deve camminare, con passo attento e con piena consapevolezza delle responsabilità che si assumono, anche un soggetto politicamente responsabile. Quindi anche questa parte del controllo parlamentare ci sembra che assuma nell'equilibrio complessivo della legge un peso determinante. Noi pensiamo, signor Presidente, che un Paese debba soprattutto avere fiducia nei suoi apparati di sicurezza; questa è, credo, la formula che esprime correttamente il senso, l'obiettivo che una normativa generale sul punto deve cercare di perseguire. Fiducia negli apparati di sicurezza che, dobbiamo dire, è stata, anche in tempi recenti, notevolmente scossa da vicende che sono che sono state portate all'attenzione dell'opinione pubblica e che quindi sicuramente trovano in questo passaggio, in questa innovazione legislativa la possibilità, l'occasione di rinsaldare un rapporto che ha avuto elementi di tensione. Da questo punto di vista riteniamo opportuna l'adozione di questo testo legislativo, di questa riforma. La riteniamo complessivamente accettabile e, come dicevo, da valutare nell'insieme positivamente e per questo voteremo a favore del

Signor Presidente, il provvedimento in esame costituisce certamente un passo in avanti, non conclusivo: la legge è complessa, il suo motore sarà costituito dai regolamenti. Si poteva fare meglio dal punto di vista dell'impostazione strutturale. Questa è una via intermedia tra il sistema che stiamo per lasciare alle nostre spalle, quello della duplicità dei Servizi con una segreteria di coordinamento e quello dell'unicità che, a mio modesto avviso, avrebbe consentito una maggiore efficacia operativa. La prima sfida che la nuova struttura dovrà affrontare sarà proprio quella di garantire un raccordo effettivo e penetrante tra due Servizi che restano, nonostante le denominazioni, distinti. Un'altra sfida che interessa entrambi i Servizi, oltre che l'organismo di raccordo, sarà quella di una seria ripartizione di competenze, senza sovrapposizioni ma anche senza lacune. Si poteva fare di più sulle garanzie funzionali. Troppi limiti, probabilmente esito delle polemiche degli ultimi anni e degli ultimi mesi, che hanno condizionato e fatto estremamente circoscrivere ciò che può essere autorizzato dal vertice di Governo con un meccanismo che, per certi snodi, appare troppo macchinoso. La trasparenza poteva essere resa meglio nel reclutamento e nella gestione del personale e il ruolo della scuola, che ha di positivo di essere unica, incontra ancora eccessiva timidezza nei risvolti che può avere per l'avvio all'attività operativa, che non appare totalmente obbligatorio per tutti coloro che entrano nei Servizi. Da ultimo, tra le riserve, evidenzio un ruolo ancora limitato dell'organismo parlamentare di controllo. Abbiamo avuto modo, signor Presidente, di cogliere insieme, negli organismi di raccordo di una grande democrazia, qual è quella degli Stati Uniti d'America, il fastidio e il disagio dei Servizi che si sentono sottoposti a controllo, il che è un dato positivo, perché significa che il Parlamento il controllo lo esercita e in modo penetrante. Non aver fornito il COPACO di tutti gli strumenti di cui poteva disporre credo che renderà questo controllo più problematico. Nonostante ciò e con queste perplessità, Alleanza Nazionale non farà mancare il proprio voto favorevole al provvedimento, pur essendo gelosa delle proposte che ha presentato e che sono confluite in questo testo comune, presentate dal presidente Ramponi, forte anche della sua qualificata esperienza professionale, e da chi sta parlando in questo momento. In trent'anni è cambiato il mondo, non solo per quello che è accaduto attorno al 1989 ma anche e soprattutto per l'11 settembre; non sono cambiati in Italia, a differenza di quello che è avvenuto in altri Paesi, gli assetti dei Servizi. Oggi registriamo questo passo in avanti, al quale diamo questa fiducia con perplessità, con riserva. Ci auguriamo - lo auguriamo a coloro che sono al lavoro in questa direzione - che i regolamenti siano scritti nel modo chiaro e più omogeneo possibile, che vi sia un coordinamento effettivo tra il lavoro di coloro che stanno stendendo i Servizi, che le risorse - così come è riportato nell'ordine del giorno che il Governo, sia pure con delle limature, ha accolto - siano finalmente adeguate, perché non è possibile che i Servizi operino per il 2007 con la metà delle risorse del 2006; che cessi questo alone di sospetto nei confronti delle strutture nel loro insieme, che non possono essere indebitamente giudicate in modo negativo per comportamenti eventualmente illeciti di singoli appartenenti ai Servizi stessi. L'approvazione di questa legge è anche l'occasione per esprimere gratitudine a tutti coloro che nei Servizi hanno ben operato fino a questo momento, garantendo un'adeguata prevenzione dai rischi per la sicurezza dell'Italia. *(Applausi

la base organica portante: prima essa era divisa tra esteri e controspionaggio, che facevano riferimento alla Difesa, l'ex SISMI, e l'altro Servizio che faceva perno sull'Interno, sull'Interno, il SISDE; adesso nella sostanza le due Agenzie ricalcano l'incardinamento precedente. Non vi è dubbio che tutto quello che è successo anche in tempi abbastanza recenti

condivisibile per due motivi. Innanzitutto vi è un maggior controllo governativo sui Servizi, ma - c'è anche un contraltare - anche maggiori poteri ispettivi da parte del Parlamento sulle attività sia governative che dei Servizi. Non era male per noi nemmeno quel tentativo che si esperì sotto il Governo Berlusconi; peccato che ci fu un'*impasse* perché anche in quel caso due Ministri, della difesa

Condividiamo l'impostazione delle due agenzie che rispondono direttamente al Presidente del Consiglio, il quale potrebbe, se lo richiede, trovare anche una forma di autorità delegata, un Ministro, al quale

subire questa procedura speciale secondo la quale per 15 anni non dovrebbero essere resi pubblici, salvo la necessità di prorogare per altri 15 anni questa copertura.

non finiscano sui giornali perché, con tutta la buona volontà, ciò che è accaduto, il fatto che un magistrato abbia messo in fila una serie di agenti segreti che operano in ambienti estremamente a rischio, è stato un po'come

dovessero verificare dei fatti e le stesse Regioni fossero minacciate nel contingente. Spiace, perché sarebbe stata l'occasione per un buon coinvolgimento dei territori nell'attività complessiva dei Servizi di sicurezza di questo Paese. Per tutto il resto la Lega esprime parere favorevole.

pervenire ad un testo che sicuramente razionalizza e rende più efficaci quegli strumenti fondamentali per la sicurezza dello Stato che sono, per l'appunto, i Servizi di sicurezza. Il provvedimento offrirà strumenti migliori sia di azione, sia di controllo, sia di tutela rispetto a queste attività. Formulo l'auspicio che, una volta approvato il provvedimento, vi sia da tutte le parti in causa un senso di responsabilità, un senso di responsabilità, che è doveroso quando si tratta - come in questo caso - di tutelare la sicurezza dello Stato, dei cittadini e dunque di

al quale fanno capo parecchie responsabilità; vi sarà bisogno del senso di responsabilità della direzione e di tutto il personale dei Servizi di sicurezza, dell'organo dell'organo parlamentare di controllo, delle Forze di polizia e della magistratura, che saranno chiamate ad una leale e positiva collaborazione. Non si tratta di un un campo di scontro per far avanzare la propria parte politica, ma si tratta di tutelare la sicurezza dei cittadini e dello Stato. È un settore importante della nostra vita pubblica e quotidiana, che giustamente ha trovato l'accordo qui, in Parlamento. L'importante è che l'accordo volto al bene pubblico continui nell'applicazione di questa legge: sarà molto difficile, ma ancora più importante.

Presidente, mio malgrado, devo differenziare il mio voto da quello del mio Gruppo. Sulla base di una conoscenza non superficiale e a tratti anche dolorosa dei fatti, ho sempre sostenuto la necessità di una riforma radicale dei nostri Servizi di informazione e di sicurezza che ci portasse ad un Servizio unico impostato su due branche e sottoposto direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Ancora oggi sono convinto che in tal modo saremmo arrivati a Servizi più agili, più efficaci, meno costosi e più controllabili. Inoltre, nella concreta attuazione di una riforma siffatta, avremmo potuto più agevolmente rimuovere sovrastrutture, incrostazioni, ruggini che si sono accumulate negli anni e che purtroppo sono state causa di inconvenienti diversi e anche di gravi rischi. Riconosco che il testo che ci accingiamo a votare contiene significative e positive innovazioni,

le ragioni che ho appena evocato e un dovere evidente di coerenza mi impediscono di esprimere un voto favorevole. Pertanto, non parteciperò alla votazione.

di sei anni fa, il Comitato parlamentare di controllo sui Servizi di informazione e sicurezza del nostro Paese approvò, rapidamente e all'unanimità, un documento in cui venivano tracciate le linee di quella che fu ritenuta immediatamente una riforma indispensabile. Rispetto al nuovo terrorismo internazionale,

Appariva ormai chiaro al nostro Paese (ma lo era, per la verità, già nella legislatura precedente inaugurata nel 1996) che lo strumento della *intelligence* italiana mostrava tutto il peso degli anni.

era radicalmente e profondamente mutato. Occorreva, da un canto, dare più efficacia all'azione dell'*intelligence* e, contestualmente, alzare la capacità di controllo, anzitutto parlamentare, sul lavoro di questa.

servizio militare e civile, ripartizione chiaramente frutto del passato contesto. È eliminata la doppia dipendenza dal Ministero della difesa e da quello dell'interno e, sostanzialmente, la responsabilità è affidata alla Presidenza del Consiglio. Sono introdotte le garanzie funzionali, così fortemente richieste dagli operatori, che nel passato sistema erano di fatto attuate con lo strumento improprio della opposizione del segreto di Stato per impedire che operatori della *intelligence* potessero essere condannati per avere espletato funzioni comunque attinenti al loro servizio. È introdotto un più efficace controllo parlamentare, e noi siamo asso0lutamente convinti che, per evitare deviazioni e usi impropri in una materia così delicata, lo strumento più efficace sia proprio il controllo parlamentare. È, infine, limitata nel tempo la durata del segreto di Stato, e questo consentirà al nostro Paese, anche rapidamente, di conoscere la verità su vicende alle quali non è più necessario opporre tale segreto.

sarebbe stato possibile immaginare e forse fra qualche tempo sarà possibile compiere un ulteriore passo nella razionalizzazione dell'*intelligence*; si potrà arrivare, io penso, ad un Servizio unico, con diverse agenzie specializzate al proprio interno.

il particolare valore assunto, anche in un clima di forte contrapposizione tra maggioranza e opposizione, dalla circostanza che su questa legge tanto alla Camera quanto al Senato sia possibile trovare le ragioni di un bipolarismo intelligente e temperato,

di solito, il Governo fornisce delle risposte bibliche. È un'interrogazione che riguarda la banca Italease. Oggi tutti i giornali (ormai da una settimana tutti i giorni) illustrano una situazione inquietante per quanto riguarda questa banca. Addirittura, ci informano che tutto il consiglio di amministrazione è stato sciolto dalla Banca d'Italia, un consiglio di amministrazione dove siedono i più importanti banchieri d'Italia. Poiché in questa interrogazione sollecitavo il Governo affinché rendesse noti i suoi intendimenti e lo stato dell'arte, ora credo sia più che mai doveroso sollecitare una risposta per gli elementi e le notizie inquietanti che quotidianamente ci vengono forniti